rendere una comunicazione alla Presidenza e all'Assemblea. Ieri è successo, in provincia di Agrigento, un fatto gravissimo: è stata data alle fiamme la casa famiglia del sindaco attualmente in carica della città di Licata. È un fatto odioso, che assume ancora maggior significato perché a Licata,

Si sta facendo questo in ottemperanza a un protocollo di intesa tra la procura della Repubblica di Agrigento, il Comune di Licata e altre amministrazioni, firmato il 7 ottobre del 2015. di un atto particolarmente grave, che fa seguito anche ad altri atti intimidatori nei confronti delle imprese che stanno svolgendo questo genere di attività e, tra l'altro, lo stesso sindaco è stato bersaglio di una intimidazione fisica non più tardi del mese di febbraio del 2016.

nella giornata di ieri erano già presenti il prefetto e il questore e oggi anche il Ministro dell'interno si è recato in visita alla città di Licata. Un problema di questo genere non può vedere distante o distratto il Parlamento. Occorre, a mio avviso, trovare nuove formule che possano mettere al sicuro l'incolumità degli amministratori locali, magari dando compiti e funzioni ad alcuni istituti e ad altri organismi,

Presidente, nel ribadire la piena solidarietà nei confronti di questo sindaco, che è stato vigliaccamente e vilmente offeso, non solo nella sua persona, ma anche nelle cose materiali, solo ed esclusivamente per aver fatto rispettare la legge,

che stanno assistendo ai nostri lavori, ai quali purtroppo devo comunicare che la seduta è sospesa fino alle ore 17,15.

**Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016

**Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015

e sono stati accantonati

volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare. volte a prevedere l'inserimento in etichetta, sotto la responsabilità del produttore o del confezionatore, del termine minimo di conservazione entro il quale gli olî di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta qualora il 100 per cento degli olî proviene da tale raccolta.

a questa proposta di stralcio dopo il lungo dibattito che si è svolto nell'ultima seduta sull'articolo 3 così come era stato proposto dal Governo, a seguito della presentazione di molti emendamenti soppressivi di quell'articolo e di un'ampia e dichiarata volontà da parte dell'Assemblea di volerne approvare la soppressione. Ora, non starò a discettare sul fatto che la proposta di stralcio potrebbe, anche ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, avere una controindicazione; sono stati espressi pareri diversi in Commissione bilancio, la Commissione ha votato sul nulla osta e non tornerò sull'argomento. Ma, dal punto di vista politico, intendo rivolgermi al Governo, che si apprestava a proporre una norma al solo fine di evitare una possibile procedura di infrazione; una norma che, a detta di tutti gli intervenuti la volta scorsa e di tutti noi che ne abbiamo poi condiviso gli argomenti, sarebbe stata fortemente penalizzante per il comparto agricolo e, in particolare, olivicolo del Paese.

quello di ricercare soluzioni per evitare che la normativa europea penalizzi i nostri prodotti e per evitare che noi, difendendo i nostri prodotti, possiamo eventualmente incorrere in una procedura di infrazione, dalla quale il Governo deve difendere il Paese e i suoi produttori.

sarebbe non solo riduttivo, ma anche una cartina di tornasole della volontà del Governo di non evidenziare le sue contraddizioni o le contraddizioni tra il Governo e l'Assemblea e, quindi, di non voler dare voce al Parlamento nel bocciare anche alcune proposte del Governo. Quindi, ripeto, noi e soprattutto il Governo dobbiamo trarre le conclusioni politiche del punto di mediazione al quale si è giunti. Il Parlamento non accettava quella norma perché riteneva prioritario l'interesse dei produttori italiani rispetto ad una possibile

d'anni. Vi è tutto il tempo, quindi, perché il Governo si adoperi in sede europea perché le ragioni dei nostri produttori prevalgano sulla solita normativa un po' burocratica e un po' farraginosa dell'Unione europea che poi porta anche alla procedura di infrazione.

che tale stralcio sia un ripensamento da parte del Governo e una dichiarazione di impegno a far sì che non vi sia la necessità di approvare in futuro una norma simile, e dunque che quello di oggi non sia solo un differimento, ma un impegno a far sì che la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia venga bloccata, rispettando prioritariamente gli interessi dei nostri produttori, in questo caso quelli del settore olivicolo in modo particolare.

È stata una vittoria dell'Assemblea, ma anche del Governo che ha saputo accettare le nostre proposte.

Signor Presidente, il sottosegretario Gozi sa che una delle caratteristiche fondamentali dell'intelligenza, specie dell'intelligenza umana, è la duttilità. Questo è un caso in cui la duttilità dei comportamenti ha avuto la meglio sulla rigidità delle questioni e dei principi.

Prima o poi, noi dobbiamo intenderci su una serie di questioni. C'è infatti la questione fondamentale della tutela del *made in Italy* e c'è la questione fondamentale della tutela dei produttori e dei diritti dei consumatori.

interessi e queste posizioni, perché la somma di queste posizioni e di questi interessi costituisce, in un *unicum*, l'agroalimentare che fa grande il nostro Paese e che fa grande soprattutto il *made in Italy*. Quindi, nell'esprimere la soddisfazione del Gruppo di Area Popolare, lancio allo stesso tempo un invito al Governo ad aprire un dibattito in Parlamento su queste questioni, in maniera tale da intenderci una volta per tutte. [DE

Grazie,

all'articolo 3, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge, che sarà immediatamente deferito alla competente Commissione parlamentare.

il Governo accoglie convintamente l'ordine del giorno presentato dal senatore Ruta, che ringrazio per questo. Tanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quanto quello della giustizia ritengono necessario ed urgente il riordino delle norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (l'agropirateria, la contraffazione, le agromafie

che ha concluso i suoi lavori lo scorso mese di dicembre. Il Governo è quindi intenzionato, facendo tesoro delle proposte emerse in tale commissione, a presentare un apposito disegno di legge entro la pausa estiva.

che erano inammissibili, almeno in questo provvedimento, anche perché riguardavano una fattispecie che tendeva a contrastare alcuni comportamenti, senza avere nulla a che vedere con il provvedimento di cui stiamo parlando.

ora che tale articolo è stato stralciato, su proposta del Governo, condividendo il percorso di andare insieme nella direzione della salvaguardia di tutte le nostre filiere agroalimentari,

Presidente, prendo la parola sugli emendamenti 18.200 e 18.201 di cui sono firmatario: si tratta di due emendamenti che hanno lo scopo di portare dal 50 all'80 per cento il regime di forfetizzazione previsto dalla *tonnage tax* (istituto tributario introdotto nel nostro ordinamento nel 2003),

Quel nuovo regime è stato particolarmente utile, direi anzi provvidenziale, perché ha consentito uno sviluppo, che prima non c'era, della marineria italiana tanto con il registro nazionale che con quello internazionale. Oggi attraversiamo una le compagnie di *shipping* che usufruiscono di questa forfetizzazione hanno raggiunto il tetto del 50 per continuare a crescere, così come noi tutti auspichiamo, assicurando prodotto interno lordo al nostro Paese e anche gettito tributario, hanno la necessità di godere di una forfetizzazione fino all'80 esattamente come accade nella stragrande maggioranza dei Paesi comunitari, senza menzionare il caso di Malta che arriva al 100 per cento. Questo è la finalità degli emendamenti.

emendamento - propone un procedimento di delega complessiva molto ampia al Governo, nella quale - ma chiedo conferma di questa disponibilità e volontà proprio ai banchi del Governo

Questo è il prima problema che pongo, annunciando altresì che, in virtù di questa delega, provvedo al ritiro degli emendamenti 18.200 e 18.201. Come dicevo, vorrei anche esprimere la

che quel comma non è la definizione di un principio delega in base al quale il Governo provvederà alla definizione e approvazione di un provvedimento delegato. Qui siamo già

che utilizzano - attenzione - esclusivamente personale italiano o comunitario. Lo dico in altri termini:

con passaporto canadese - perderebbe tutti i benefici tributari, contributivi, che la Repubblica gli assegna. Io suggerirei prudenza al Governo. Concludo con una notazione di carattere squisitamente politico. Noi abbiamo assistito, nel corso dei mesi passati, ad una conflittualità decisamente acuta tra armatori. Il mondo armatoriale italiano è connotato da una fortissima conflittualità a cui si riferisce anche questa normazione. A me pare che il Governo farebbe bene ad avere un profilo politico che smorzi i conflitti e non che li attizzi. Credo che questa normazione finirà per attizzare i conflitti, e mi pare un profilo politico sbagliato. Aggiungo anche che nella conflittualità che - Dio non voglia - potrebbe essere attizzata da queste norme, potremmo anche arrivare a mettere in discussione il quadro delle norme che favoriscono la continuità territoriale con la Sardegna. Questo mi sembrerebbe un autogol. Sulla base di tutte queste considerazioni, invito a riconsiderare attentamente le norme che qui ci vengono

ovviamente d'accordo sulla necessità di rivedere con una delega al Governo tutte le normative che riguardano la materia degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi delle imprese marittime,

Di fatto c'è un duopolio rispetto al quale, con una norma siffatta, il Parlamento sceglierebbe uno dei due soggetti in maniera evidente e senza passare attraverso la Commissione competente. Mi è stato detto che questa norma favorirebbe la continuità marittima in Sardegna. A tal proposito segnalo che la continuità marittima in Sardegna non funzionava con un solo soggetto; oggi inizia ad essere un sistema più competitivo perché ci sono almeno due soggetti che competono. Sarebbe bene favorirne ancora di più, anche perché i prezzi per connettersi alla Sardegna nel periodo turistico o per il

un voto di astensione sarebbe il minimo di fronte al mantenimento della proposta emendativa

da mettere insieme diverse sensibilità e questioni sia di natura economica, che di principio. parere, è importante il riferimento al rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea previsto dal comma 10-*ter,* che regge complessivamente l'intero articolo e, quindi, anche i principi in materia di lavoro e discriminazione.

29.300 e parere contrario

non soltanto coloro che hanno un limite reddituale, possano beneficiare di questo indennizzo.

Siamo assolutamente sensibili alle istanze da lei sollevate. Questo è un primo passo nella risoluzione di una questione che per il Governo è prioritaria. Ci impegniamo a lavorare per raggiungere molti, se non tutti, gli obiettivi perseguiti dalla senatrice Bencini con questo emendamento, che

patrocinio a spese dello Stato; *b)* che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

della tutela dei nostri prodotti agricoli. Non c'è la volontà di andare avanti; delle etichettature di sicurezza non si parla assolutamente, forse per favorire - lo devo dire - *lobby* italiane.

Aula. Sinceramente non si può aver fiducia del modo di operare del Governo. Viene meno ogni speranza; c'è una latitanza rispetto ai problemi perché forse non c'è il coraggio né la volontà di affrontarli. Pertanto il nostro voto resta di astensione, ma per quanto ci riguarda è già uno sforzo rispetto al nulla che avete manifestato anche in questa occasione.

arriva da quell'Europa che tutti conosciamo, quella dei burocrati; arriva da quell'Europa che ci impone le sue scelte alle quali noi ci dobbiamo adeguare. Noi l'abbiamo detto in più di un'occasione: stare in Europa a queste condizioni non ci piace, non ci è mai piaciuto e non piace a tutti gli operatori che, grazie a questo provvedimento, dovranno subire ulteriori danni. Come abbiamo detto in più di un'occasione, il voto della Lega sarà quindi contrario. Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, debbo dire che è davvero imbarazzante la la discussione che si è tenuta a proposito della legge comunitaria; è stata imbarazzante sin dai primi passi che ha mosso in Commissione,

non si presenta in Parlamento con una visione composita, chiara, definita; un Governo che, di converso, ha assolutamente bisogno di aggiornare quasi quotidianamente le proprie posizioni, su una norma che è di carattere fondamentale,

Non ci piace quando il Sottosegretario limita la propria disamina di carattere politico-istituzionale ai confronti con il passato; preferiremmo che il Sottosegretario avesse l'onestà intellettuale di fare il confronto con se stesso e con l'azione del suo stesso Governo.

Preferiremmo che il Governo facesse un'analisi complessiva di ciò che sta facendo e di ciò che vuole realizzare in tema di politiche agricole.

Sapete che una singola normativa non solo non tutela, ma "mette sotto scopa", cioè a disagio, le produzioni agricole dei nostri territori quindi di riflesso i nostri mercati subiscono una concorrenza dei prezzi assolutamente sleale? I nostri produttori subiscono cioè una concorrenza assolutamente sleale, perché i prodotti provenienti

A fronte di questo, però, non solo non si aprono tavoli di crisi, non solo non si assumono provvedimenti eccezionali come la moratoria sulle cartelle esattoriali,

delle normative europee si adotta una postura supina rispetto a determinazioni che sappiamo ci danneggeranno moltissimo.

di qualunque violenza è sempre vittima di reato. Siamo solo noi che ancora ci ostiniamo a dividere le vittime di reato e a riconoscere tutela giuridica solo a coloro che siano vittime di associazione mafiosa o di usura. È una norma di assoluta civiltà e di giustizia che uno Stato deve riuscire a garantire a tutti i cittadini; ne va della credibilità e della serietà dello Stato.

voglio solo denunciare il voto favorevole o contrario sul singolo emendamento - che poi ha determinato lo stralcio dell'altra norma,

cuore i problemi che sono sulla carne viva dei cittadini (come quelli delle vittime di reato e della nostra agricoltura), ma non ha neanche un disegno organico su come superare queste criticità. non ha un'idea di cosa viva il cittadino che sia vittima di un reato, di quale devastazione viva nel proprio nucleo familiare, nella propria azienda economica. Cosa fa questo Governo oggi, 10 maggio? Ci propone ancora una volta di rinviare questi problemi, che sono sulla carne viva del nostro popolo, le disgrazie che vengono avvertite in maniera più dura e cruenta.

che in una materia come la legge europea, su cui non ci siamo mai strettamente schierati tra maggioranza e opposizione, perché è un tema su cui abbiamo cercato di lavorare

europea, ma sappia anche proporre alla comunità europea una posizione italiana e, una volta tanto, mostri che le posizioni italiane vengono recepite a livello europeo (e non che, in maniera supina, vengono recepite le posizioni europee sul territorio italiano).

*(AL-A (MpA))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, con la legge europea 2015 si pone rimedio a numerose situazioni di infrazione consentendo all'Italia di compiere interventi normativi utili a introdurre disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per attuare o applicare correttamente gli atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Sappiamo come sempre di più, negli anni scorsi, il nostro Paese - soprattutto su alcune tematiche, per esempio quelle di carattere ambientale - sia stato caratterizzato da disomogeneità nell'attuazione puntuale della normativa europea. A giudizio del nostro Gruppo, il Governo ha impresso un cambio di marcia apprezzabile riducendo il numero delle infrazioni a carico dell'Italia, come evidenziato ieri dal relatore, al minimo storico. Certo, molto ancora resta da fare perché a carico del nostro Paese restano ancora 80 procedure; ma il cammino avviato - ci sembra - va nella giusta direzione. È inoltre da evidenziare che nei giorni scorsi è stata trasmessa al Senato, dopo l'approvazione della Camera avvenuta il 27 aprile, la legge di delegazione europea, il provvedimento che contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento degli atti dell'Unione europea (ad esempio direttive dell'Unione o decisioni quadro) che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali. Nello specifico del testo al nostro esame, apprezziamo in particolare alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame nella Commissione politiche dell'Unione europea. Faccio tre riferimenti in particolare, accompagnati da poche parole di spiegazione: all'articolo 5, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Questa è una norma a tutela dei consumatori, per esempio con riferimento al detergente liquido per bucato contenuto in un imballaggio solubile monouso e destinato alla vendita al pubblico. all'articolo 20 che pone fine a una procedura d'infrazione contro l'Italia in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e che recepisce nell'ordinamento la direttiva sul trattamento fiscale di dette società. Giudichiamo in modo positivo che vengano eliminati dei vantaggi fiscali per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale degli utili distribuiti nelle legislazioni degli Stati membri. l'articolo 29 che riconosce, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di una norma che consente di combattere il cosiddetto caporalato, un fenomeno grave e inaccettabile che caratterizza ancora molte realtà agricole del nostro Paese.

come ampiamente è emerso in questo dibattito parlamentare, e bene ha fatto il Governo a recepire anche le istanze pervenute dal nostro Gruppo parlamentare per quanto riguarda l'articolo 3, che è stato in effetti ritirato. Sulla base delle ragioni sopra esposte, sia di contesto generale che in riferimento al contenuto del provvedimento in esame, dichiaro a nome del Gruppo parlamentare AL-A il voto favorevole alla legge europea 2015-2016. Altrettanto faccio per le risoluzioni trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione europea, evidenziando - nel contesto storico spesse volte drammatico che stiamo che stiamo vivendo nel Mediterraneo e in terre vicine come il Nord Africa e il Medio Oriente - i temi dell'immigrazione, della lotta al terrorismo e della risoluzione dei conflitti oggi in corso in realtà come la Siria e la Terra Santa. Su questi *dossier*, come il nostro Gruppo ha avuto modo di affermare ancora di recente in quest'Aula durante le ultime informative del Ministro degli esteri e nel *question time* della scorsa settimana sulla Siria, è necessario un impegno forte e reale dell'Europa, certamente con il sostegno deciso da parte dell'Italia che ha il dovere di giocare in pieno il proprio ruolo di Paese guida nel cuore del Mediterraneo.

per andare un po' oltre la mera illustrazione delle ragioni e delle motivazioni che portano il mio Gruppo ad astenersi dal voto sui provvedimenti Voglio infatti provare a lanciare un ulteriore SOS per sottolineare quel dato ormai macroscopico e preoccupante che senza un radicale cambio di marcia continuerà a sconquassare e dilaniare gli interessi del nostro Paese in Europa. Infatti anche oggi quanto verrà approvato - perché credo verrà approvato - di fatto non andrà ad aggredire adeguatamente ed efficacemente la radice e la ragione di cui il provvedimento in esame è un mero effetto e che è possibile riassumere nel vuoto di politica che l'Italia sconta da troppi anni in Europa. Credo sia ineludibile avviare una discussione profonda, un'analisi critica e chirurgica sulla tipologia e la graduazione del rapporto tra il Parlamento nazionale, i rappresentati nazionali nel Parlamento europeo e gli organi di decisione dell'Unione stessa. La discussione congiunta della legge europea, da un lato e, delle risoluzioni sulle priorità dell'Unione per il 2016 e sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015, dall'altro, ci palesa in modo plastico questa assenza di un valido, capace ed efficace interlocutore della politica e delle politiche italiane a livello europeo, di una valida ed efficace rappresentanza a difesa dei nostri interessi nazionali. Oggi infatti abbiamo rischiato - ed abbiamo evitato questo rischio solo in calcio d'angolo - due diversi tipi di provvedimenti, due iniziative distinte, ma che potevano rappresentare l'*ex ante* e l'*ex post* di questa grave assenza. Da un lato infatti, con la risoluzione n. 56, voteremo certamente un'agenda dei sogni, con la quale impegniamo il Governo ad adoperarsi in sede europea per scongiurare la Brexit, a far valere i principi di solidarietà e di leale collaborazione nella drammatica gestione dell'emergenza dei flussi migratori, a rivedere il superato Trattato di Dublino, a far rispettare i principi e valori della nostra Costituzione (quale?) nei contenuti del TTIP, a contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane e, così a seguire, molti altri nobili impegni dichiarati. Ma allo stesso tempo, dall'altra parte, stavamo per approvare la legge europea 2015, che altro non è e che altro non sarebbe potuta essere che una sorta di norma-patteggiamento, una norma-sanatoria dei contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello e quello europeo (ma non nel nostro interesse). Una norma che è difficile da mandar giù - e sarebbe stata ancor più difficile da mandar giù, se non ci fosse stato l'intervento di

trova la propria approvazione solo perché consente alle casse dello Stato di evitare di incorrere in sanzioni che producono effetti negativi sulla finanza pubblica. Anche quest'anno, quindi, in nome di una soluzione veloce dei casi di pre-infrazione, rischiavamo di immolare sull'altare delle direttive europee alcune produzioni agricole italiane di particolare rilievo qualitativo e identitario. Purtroppo è qui che si riscontra e si sconta l'assenza di un vero peso politico del nostro Paese in Europa, che - sia ben chiaro - non può continuare ad essere barattato con il risultato, positivo ma troppo modesto, di una riduzione del numero delle infrazioni dell'Italia, anche perché le ricadute di questo saldo e di questa chiusura delle infrazioni si abbattono sempre e si schiantano, come vere e proprie mannaie, su un comparto produttivo strategico, qual è appunto quello agroalimentare. L'articolo 1 di questo provvedimento è - consentitemi - quasi un epitaffio sulla produzione italiana e soprattutto sulla produzione italiana di qualità dell'olio di oliva. Insomma questa Europa, dopo aver invaso e dopato il mercato con l'olio tunisino, dopo averci regalato disciplinari insopportabili come le indicazioni geografiche protette, adesso ci obbliga ad abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. Questa misura chiaramente non ha ricadute dirette nei confronti di prodotti e produzioni non di qualità; ma in Italia, dove le produzioni di qualità abbondano, prevedere una misura del genere, genere, abbandonarsi ad accettare una misura del genere, segna un danno di assoluta rilevanza. E allora ecco che lo stralcio dell'articolo 3 è certamente una nota positiva è una scelta saggia; ma è una riduzione del danno, perché ci espone comunque ad una procedura di infrazione che non dovrebbe nemmeno aver motivo di esistere.

che l'auspicato rafforzamento e consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, previsto nella risoluzione n. 59, diventa una necessità non più rinviabile rinviabile e impellente, perché occorre coordinare la partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Europa, nella fase sia ascendente che discendente della normativa europea, ed occorre essere preparati nell'approccio della risoluzione dei casi di contenzioso e precontenzioso. Occorre istituire una vera e propria *task force,* per rappresentare e difendere le produzioni e i territori italiani. Si tratta - ed è bene ricordarlo sempre - di andare a difendere principi che si trovano implicitamente espressi nell'idea stessa dell'unione dei popoli europei, dove il rispetto e la tutela delle differenze, delle peculiarità e delle tipicità costituiscono una declinazione portante e fondante dell'idea stessa di Europa. L'invito e l'auspicio che faccio, anche qui oggi, è quello che il Governo, nei diversi tavoli negoziali, mantenga con fermezza la salvaguardia degli interessi italiani e che non deleghi sempre rappresentanti distratti; ma sono altrettanto consapevole che, al Parlamento di Bruxelles, scontiamo l'assenza di un fronte politico unito, capace realmente di coordinare e strutturare la difesa e la tutela dei nostri interessi, anche attraverso delle alleanze strategiche con gli altri Paesi. Alla luce di queste considerazioni, in coerenza con i voti espressi gli scorsi anni su tali prassi normative, che non sembrano cambiare, e per l'immancabile senso di responsabilità, ribadisco l'astensione squisitamente e prettamente politica del Gruppo su questo provvedimento, che ha purtroppo una natura troppo e solo burocratica.

siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo. Mi preme sottolineare come, grazie all'attività parlamentare, i provvedimenti di tale natura siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento degli obblighi comunitari, la qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia. La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva dalla natura eterogenea della legge europea, in cui devono confluire tutte le norme dirette a sanare eventuali contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, derivanti da inadempimenti o violazioni delle norme dell'Unione. tali contrasti legislativi devono essere oggetto di specifico rilievo nell'ambito di procedure di contenzioso o precontenzioso europeo, ovvero devono essere oggetto di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione, casi EU Pilot o procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato. Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Governo riferisce che con le ultime leggi europee è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione EU Pilot e delle procedure di infrazione. Al 28 aprile 2016, il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese risulta pari a 80, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Già il precedente dato di gennaio, secondo le dichiarazioni del sottosegretario Gozi del 19 febbraio 2016, rappresentava il numero più basso degli ultimi vent'anni e l'Italia si trova ora tra i Paesi che, in termini relativi, è migliorato di più in questo ambito. Il disegno di legge è composto da 38 articoli suddivisi in 8 capi, concernenti i seguenti settori: libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, giustizia e sicurezza, fiscalità, dogane e aiuti di Stato, trasporti, ambiente, energia. 22 articoli sono volti a chiudere procedure d'infrazione e casi EU Pilot e a sanare procedure in materia di aiuti di Stato; 16 articoli introducono modifiche alla normativa interna per prevenire procedure d'infrazione. Tra le norme del testo si segnalano, in particolare, le seguenti: l'articolo 6, volto a sanare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) l'obbligo di avere la sede legale in Italia, prevede, a modifica dell'articolo 64 del DPR 207/2010, che tali società abbiano in Italia una sede qualsiasi anche solo operativa. L'articolo 28 interviene sul terzo pacchetto energia la procedura d'infrazione UE per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e 2009/73/UE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia e del gas naturale. In particolare, viene modificato l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011 con la previsione che il Ministero dello sviluppo economico possa fornire indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi (e non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri dell'Unione europea). Viene, altresì, modificato l'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011 per dare la possibilità ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE. Viene, inoltre, modificato l'articolo 45 sul potere sanzionatorio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'articolo 35 è volto a modificare la normativa relativamente alla figura del segretario generale del Comitato interministeriale per gli affari europei. L'articolo 36 è volto a sanare una procedura d'infrazione sulle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato di cui alla legge n. In particolare, viene previsto che le amministrazioni centrali e territoriali, che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongano la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche europee) attraverso il sistema di notificazione elettronica, anziché provvedere direttamente all'inoltro alla Commissione europea. Quest'ultima effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall'articolo 3 del regolamento CE n. 794/2004). Queste sono solo alcune delle norme in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, del nostro tessuto sociale ed economico, seppure nel quadro di un interesse più generale che è quello di un'Unione europea coesa e funzionale. Pertanto, Area Popolare voterà convintamente a favore di questo provvedimento con la convinzione che l'Italia possa giocare un ruolo da protagonista nel futuro dell'Europa unita.

molto l'amaro in bocca in tutta questa legge europea è il famoso articolo sul gioco *on line* che non riusciamo proprio ad accettare. Quindi, già dà adesso preannuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle perché, come sempre, infilate cose assolutamente ignobili in un contesto che avrebbe una sua dignità

dal canto suo, per esprimersi in maniera intelligente, dovrebbe avere piena contezza di tutti i documenti che riguardano la fase ascendente della normativa europea. Mi trovo qui, ancora una volta, a ricordare al sottosegretario Gozi che ho presentato un'interrogazione, alla quale non mi ha risposto, a parte qualche vaga risposta, ma priva

di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, nonché i documenti di consultazione predisposti dalla Commissione europea (quali Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni), vengano trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei - purtroppo è stato abolito, ma Moavero in qualche modo ci aiutava in questa fase ascendente e, quindi, sentiamo la mancanza di un Ministro per gli affari europei - accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza

che descrivono quello che la Commissione europea ci chiede, in modo che poi andiamo sia dal legislativo sia da Coldiretti, ovvero da tutte le associazioni di categoria, a dire come rispondiamo a quel caso EU Pilot, visto che la Commissione europea ci ha dato quel foglietto.

e portatrici di effetti caratterizzati da diversa gradazione del proprio impatto sull'economia e sulla vita sociale. Se è vero che il male si nasconde nei dettagli, è bene allora notare come il provvedimento in esame contenga in alcuni passaggi punti di grande criticità per gli interessi dell'Italia. Mi soffermo brevemente su alcuni di questi. È il caso - ad esempio - della norma riguardante l'olio d'oliva, in particolare l'extravergine, che è uno dei nostri fiori all'occhiello. Nei fatti, la Commissione europea afferma il principio secondo il quale non vi è alcuna correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della sua conservazione e noi, pedissequamente - vorrei dire supinamente - la seguiamo. presupposto incide fortemente su ciò che rappresenta, invece, il nostro invidiato *made in Italy*, che basa la commercializzazione dei propri prodotti - quindi anche dell'olio di oliva - soprattutto sulla qualità del prodotto e sulla durata della sua conservazione. conservazione. Al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione europea, vi è una correlazione diretta e immediata tra la qualità e i tempi di conservazione. Infatti, per avere un olio di qualità è necessario rispettare i tempi di conservazione e occorre che questi non siano troppo lunghi. Andando oltre il tecnicismo, bisogna inoltre ricordare quanto tale settore sia rilevante per il nostro commercio con l'estero. L'Italia è uno dei maggiori produttori di olio extravergine, riconosciuto nel mondo per le sue particolari particolari caratteristiche organolettiche. Non dimentichiamoci che, proprio pochi mesi fa, la Commissione europea ha autorizzato l'accesso al mercato dell'Unione europea, senza dazi, dell'olio tunisino: 35.000 tonnellate l'anno, in aggiunta alle 56.000 già previste. una politica europea non dico miope, ma certamente scoordinata, che penalizza i Paesi europei del Mediterraneo e, in particolare, l'Italia. Dello stesso tenore sono le norme sono le norme che riguardano il miele, che ci vedono ancora una volta subire inutili imposizioni. Nel dettaglio, si prevede l'introduzione di regole concernenti l'etichettatura del miele attraverso la dicitura: produzione della CE. Come appare evidente, del *made in Italy* non vi è cenno e, anzi, diviene del tutto ininfluente dato che i consumatori finali non conosceranno i Paesi di origine della sua produzione. si va verso un'omologazione dei prodotti e dei gusti, mentre la forza della nostra produzione è l'originalità qualitativa, frutto anche della biodiversità che caratterizza il nostro Paese. In merito al caso delle norme dell'articolo 3, oggetto di stralcio, che vietano la riproduzione sulle confezioni delle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori sui Paesi di origine dei prodotti alimentari (anche in questo caso a svantaggio della produzione italiana), il Governo, a seguito di forte pressione dell'Assemblea, ha assunto l'impegno di rendere effettiva la tutela dei prodotti italiani, a prescindere dalle imposizioni europee. E questo ci trova particolarmente d'accordo. Ulteriori punti critici riguardano gli aiuti di Stato. Con l'attuale provvedimento si prevedono una procedura unica e centralizzata di notifiche delle misure attuate dalle amministrazioni centrali e territoriali nel sostenere le imprese e una cabina di regia per la gestione dei fondi strutturali. Ciò che ci viene chiesto dall'Europa, unitamente a ciò che il Governo stesso si accinge ad attuare, creerà confusione e ulteriori danni ai produttori italiani attraverso la moltiplicazione di adempimenti di adempimenti a carico del soggetto interessato. Ulteriore esempio in questo senso è rappresentato dall'aumento dell'aliquota IVA sui preparati per risotti, che passerà dal 4 al 10 per cento. Inoltre, è prevista una maggiore tassazione sui redditi dei consorzi agrari, che sale dal 40 al 50 per cento. Non dimentichiamo poi quanto i consorzi agrari stanno attualmente pagando in termini di penalizzazione, che avrà ripercussioni sul prezzo di vendita dei prodotti e dei servizi offerti agli agricoltori, già piuttosto martoriati, distribuiti nei tanti consorzi agrari presenti in Italia. Il nostro Paese subisce già una pressione fiscale insopportabile e abbiamo visto che la riduzione fiscale ha interessato solo le imprese medio-grandi e non le piccole, che saranno gravate da questi nuovi fardelli, Il Governo dovrebbe, al contrario, impegnarsi a non accettare ulteriori aumenti di imposizione fiscale o di regole perché anche le regole inutili, che alimentano la già smisurata azione della nostra burocrazia, burocrazia, costituiscono un costo ulteriore per le aziende italiane riducendone la capacità competitiva. Faccio un'osservazione rispetto all'articolo 28, relativo a disposizioni in materia di energia: bene la previsione dell'adeguamento in merito alle nuove linee elettriche d'interconnessione, dato che le infrastrutture energetiche sono una fondamentale esigenza del sistema energetico italiano, oltre che collocate nell'ambito dello sviluppo dell'Unione europea dell'energia; bene la certificazione che qualifica i nuovi gestori dei sistemi di trasmissione. Si ritiene, però, necessario rafforzare l'obbligo dei nuovi gestori di nuovi reti di confrontarsi con l'attuale gestore del sistema di trasmissione nazionale, superando le indicazioni generiche e adeguatamente operative contenute nell'attuale formulazione dell'articolo 28, nell'intento di garantire agli operatori la certezza del quadro di riferimento. A proposito dell'argomento «regolamentazione del mercato dell'energia», persa - a nostro avviso - l'occasione per inserire esplicitamente regole utili a superare condizioni di posizione dominante nel settore della vendita di energia elettrica al fine di tutelare i consumatori nella logica del mercato funzionante e libero, in merito al qual è giunto il momento di fare chiarezza. Concludendo, dobbiamo portare in sede europea quell'autorevolezza che sta venendo progressivamente meno e difendere i nostri prodotti che rappresentano la cultura, la biodiversità e la capacità tecnologica italiana. Dobbiamo, purtroppo, prendere atto che, ogni giorno, l'Italia riduce la propria sovranità e non vede garantita la puntuale applicazione del principio di sussidiarietà, a danno di cittadini e imprese che si vedono letteralmente alluvionati da norme di recepimento incomprensibili, inapplicabili e molto spesso davvero futili, in applicazione di disposizioni assolutamente inadeguate a garantire le singolarità e le eccellenze italiane, con impatto dannosissimo sulle realtà della società italiana. Non sarà certo con ulteriori controlli e proibizioni di derivazione europea che sarà possibile rilanciare la nostra sofferente economia. Per le ragioni sinteticamente richiamate e le molte altre che i colleghi hanno evidenziato in sede di discussione generale e nella trattazione degli emendamenti, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi

del Partito Democratico voteranno a favore di questo provvedimento e lo faranno per alcune ragioni essenziali e perché vogliono cogliere lo spirito dinamico e progressivo che emerge da questa discussione dopo le diverse giornate di dibattito. Voteremo a favore perché questa legge consente di aggiornare la nostra legislazione, di armonizzare in più punti la legislazione italiana con quella europea e, al tempo stesso, di ridurre significativamente il contenzioso che abbiamo con Bruxelles, che era a un livello altissimo.

momenti di discussione. E su questo punto voglio tornare, in conclusione del mio intervento. In ogni caso, con questo provvedimento facciamo dei passi avanti. Io voglio esprimere il mio ringraziamento, ovviamente, al relatore Cociancich,

anche con i loro dettagli, talora effettivamente davvero esosi e eccessivamente puntigliosi nello specifico, sono lo specchio dei problemi dell'Europa,

Il problema è come si passa dalla giusta critica ai limiti dell'Europa (non all'Europa come progetto, ma agli

ma i vari schieramenti politici dovrebbero fare una riflessione su quanto sono riusciti essi a cambiare della situazione che hanno trovato.

A meno che non lo sia l'idea di uscire da tutto, di rovesciare il tavolo, sbattere la porta e andarsene via. Ma non vedo ancora questa come una strategia politica. Eppure, Tremonti è uomo di cultura e di grande responsabilità, che ha avuto grandi responsabilità. Io non voglio usare qui gli argomenti del sottosegretario Gozi, pur pertinenti ed efficaci sul punto. Ma, se siamo qui, è anche perché il centrodestra italiano ha usato male le sue occasioni, il suo tempo e lo spazio che ha avuto con i suoi Governi per negoziare una situazione migliore. Voglio però andare oltre questa polemica. Tutti gli schieramenti politici italiani sull'Europa hanno avuto alti e bassi. Anche il centrosinistra, che pure ha il merito dell'adesione all'euro, ha avuto le sue disattenzioni e le sue titubanze. E i nuovi movimenti, come il Movimento 5 Stelle, hanno un approccio sostanzialmente antagonista e non costruttivo. Quindi, guardiamo oltre. Io propongo che tutti insieme guardiamo oltre e costruiamo spazi e

che dice tutto ciò che andrebbe fatto ma poi, in sostanza e in pratica, non cambia nulla. Serve una critica propositiva in grado di spostare davvero le cose.

riferimento per tutti, almeno sulle grandi questioni internazionali - e l'Europa sicuramente lo è - e vediamo se i vari schieramenti riescono a trovare dei punti di sintesi.

- e questo è un punto importante - un alibi per i Governi nazionali per scaricare sulla dimensione europea tutti i problemi che si trovano davanti, né una copertura per nuovi protezionismi

ma qualche volta anche noi ci lasciamo andare a qualche istinto protezionistico, che non è esattamente la stessa cosa, giusta e doverosa, del proteggere le nostre produzioni e la nostra tradizione.

penso alla discussione che abbiamo svolto sulla mozione sul Mediterraneo, che è stata un'occasione per un confronto di ampio respiro sui temi delle relazioni della nostra economia con le economie del bacino mediterraneo nel quale viviamo.

siamo bravissimi a dire che, per risolvere il problema dell'immigrazione, la prima scelta è aiutare le popolazioni nei Paesi d'origine, ma poi,

Nel frattempo noi votiamo sì per sostenere e stimolare lo sforzo del Governo. L'Esecutivo si sta impegnando in posizioni più problematiche e critiche nei confronti dell'Europa e più decise di tanti altri Paesi europei,

Onorevoli colleghi, è stata chiesta dal senatore Cappelletti la dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1954, recante modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione. Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio. Seguirà la votazione per alzata di mano.

Signora Presidente, tempo fa, il 26 gennaio, avevo già avuto modo di segnalare a quest'Assemblea la situazione della ditta Cerpelli Pompe di Seravezza, con 30 lavoratori, all'epoca, a rischio licenziamento. Presentai un'interrogazione ai ministri Poletti e Guidi, ma, naturalmente, non ebbi risposta. Nel frattempo i 30 lavoratori sono stati licenziati. La multinazionale americana Dover, che gestiva la ex Cerpelli, con la motivazione del calo del prezzo si era rifiutata di accogliere qualsiasi proposta di riconversione o possibilità di ammortizzatori utili, almeno, a chiudere una commessa di lavoro acquisita all'inizio dell'anno. Ci furono riunioni con le amministrazioni locali, tavoli regionali, ma la risposta fu sempre irremovibile: non ci sono le condizioni lavorative per tenere in vita la Cerpelli Pompe. Oggi succede che in questo stabilimento, chiuso, ci siano strani movimenti: in pratica un via vai di lavoratori indaffarati dalla mattina alla sera.

Si sono visti lavoratori della sede di Merate in fabbrica a fare *test,* e ripeto *test*, e quindi funzioni di produzione, non di smantellamento, con punte di presenza di sette, otto lavoratori.

A questo punto chiediamo che sia fatta chiarezza. Io stessa mi ero spesa e avevo anche scritto alla Dover negli USA, ma ovviamente senza avere risposta. Ci chiediamo oggi: la ex Cerpelli Pompe sta continuando a produrre? Con quali forze lavoro? Sono state fatte particolari procedure per tutelare la sicurezza di chi sta lavorando

nel rispetto delle attuali normative. Certo sarebbe grave verificare azioni piratesche e annuncio già da ora che presenterò un'interrogazione ai Ministri di competenza. Speriamo che il nuovo titolare del Ministero dello sia meno deconcentrato della ex ministra Guidi. Insomma, i 30 licenziamenti nel territorio di Seravezza sono difficili da ricollocare; se poi fossero ingiustificati, sarebbe una beffa imperdonabile.

furono respinti da una grande forza di volontà e, da subito, si decise che bisognava andare avanti. Alla logica assistenziale di attesa di quello che lo Stato dovesse fare si antepose quella del «facciamo noi», senza aspettare, e tutti si rimboccarono le maniche. Le case da ricostruire divennero un simbolo, i paesi da riedificare così com'erano una sorta di identità collettiva, il lavoro un'opera in grado di resistere al tempo, un esempio cui ispirarsi. Oggi non ricordiamo soltanto un anniversario, ma evidenziamo come le risposte attive, rapide, efficienti ai problemi siano una forza, un'autentica risposta anche alle catastrofi naturali. Oggi celebriamo il modello Friuli, vanto del Paese, celebriamo la capacità e l'intuito di una classe politica solidale, coesa, efficiente, attiva e protesa verso la ricostruzione, ma soprattutto di una classe politica onesta. Ricordiamo tutti la splendida figura del commissario straordinario di Governo per i soccorsi e la ricostruzione, il grande Giuseppe Zamberletti, intervenuto nei giorni scorsi alle celebrazioni di Udine. I cittadini e le istituzioni del Friuli-Venezia Giulia seppero essere all'altezza di una immane sfida e non tradirono la fiducia che un grande uomo, Sandro Pertini, aveva riposto in loro, rivolgendo, in qualità di Presidente della Camera, uno storico messaggio

e concluse con un augurio ed un monito che i friulani seppero onorare fino in fondo: ricordare per prevenire e per saper gestire al meglio futuri

Concludo citando l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia nel 40° anniversario. «Appartenenza al territorio, consapevolezza della propria storia e cultura, partecipazione dal basso, orgoglio della propria autonomia, da un lato, e capacità capacità di ascolto, di guida e di solidarietà da parte dello Stato, dall'altro, hanno consentito di superare una drammatica distruzione e di porre le basi per un rilancio della convivenza civile in questa regione di incontro tra le civiltà latina, germanica e slava». Un grazie, il nostro, incondizionato a quanti indistintamente hanno lavorato con sacrificio e dedizione alla rinascita di questa terra straordinaria.